ha stabilito, in via transitoria, alcuni criteri di rideterminazione degli indici di coerenza e di normalità economica per la determinazione degli studi di settore. Ha anche

essa ha creato gravi problemi sia ai lavoratori autonomi sia ai contribuenti sia ai professionisti nella determinazione degli indici e dei parametri di settore.

Il problema riguarda essenzialmente il fatto che gli studi di settore in vigore sono fermi da molti anni e che la legge dell'anno scorso ha previsto che essi siano rivisti in quanto parametri indicativi importanti per le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Poiché però la procedura prevista per rivedere gli studi di settore (che, ripeto, erano fermi da molti anni) ha bisogno di un certo periodo di tempo, è stato fatto un accordo con i vari soggetti e le varie organizzazioni alla fine del 2006. Chiaramente i gruppi di lavoro che debbono prevedere i nuovi studi di settore hanno bisogno di un certo periodo di tempo. Per intervenire tra la vecchia vigenza degli studi di settore - ormai inadeguati perché fermi da troppo tempo - e i nuovi (che ancora non ci sono) sono stati individuati dalla legge indicatori macroeconomici che servono per individuare i criteri più aggiornati per valutare l'attività delle imprese e i problemi. Come lei sa, nel corso delle discussioni che ci sono state a questo proposito, ad esempio, è risultato evidente che vi sono aziende che detraggono il magazzino, salvo non averlo, oppure ci sono settori nei quali, se fosse vero che i prodotti sono conservati da molto tempo, ci sarebbero seri rischi per la salute dei contribuenti.

Da parte delle organizzazioni di categoria sono stati fatti osservare problemi e questioni. Non è vero, come viene detto, che non c'è stata da parte del Governo la volontà di affrontare i problemi, perché esattamente il 3 luglio scorso c'è stato un incontro durante il quale sono stati esaminati problemi e controversie che riguardavano appunto questi indicatori, ritenuti troppo grezzi e approssimativi. A questi si è fatto riferimento per arrivare ad una soluzione accolta dalle associazioni dei rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi. Si tratta di un vero e proprio protocollo d'intesa, cui hanno fatto seguito atti già in vigore o che entreranno in vigore a breve,

dovrà portare altre prove e dati in grado di dimostrare che sono stati posti in essere effettivamente comportamenti non congrui da parte del contribuente di cui si ragiona.

Naturalmente, la revisione degli studi di settore, quando verrà fatta, comporterà invece un impianto a regime secondo le modalità già note.

che a carico del contribuente c'è, per Costituzione e per legge, l'obbligo di dichiarare la verità e questo naturalmente non può mai essere dimenticato. In ogni caso, oltre alla circolare dell'Agenzia delle entrate che rende chiaro il criterio di interpretazione del ruolo degli indicatori, si è ritenuto necessario emanare anche una norma di legge. Ebbene, poiché il provvedimento all'esame del Senato - quello che va sotto il nome di IVA auto - aveva un percorso troppo lento ed era possibile affrontare con un percorso più veloce l'approvazione di una norma di legge, sono stati inseriti nel decreto-legge, che in queste ore è al vaglio della Camera attraverso il voto di fiducia, esattamente i testi che sono già stati oggetto di esame, anche se non di voto, da parte del Senato della Repubblica. Quindi, il Senato è a conoscenza di quello che sta votando la Camera. Il percorso accelerato del decreto in corso di conversione in questo momento alla Camera (la prossima settimana sarà già al Senato) consentirà di dare, anche per questa via, ai contribuenti certezza sul ruolo degli indicatori cosiddetti macroeconomici che hanno appunto il carattere di strumento per l'amministrazione, ma non hanno le caratteristiche di prova diretta a carico dei contribuenti, mentre costituiscono per l'amministrazione un elemento importante per sostenere il contraddittorio al fine della ricerca della verità in riferimento agli studi di settore. Mi permetto di dire, alla fine, che non c'è più quel clima cui si fa riferimento nell'interpellanza, perché l'ascolto che il Governo ha avuto nei confronti delle categorie che rappresentano i lavoratori autonomi e i professionisti ha consentito di individuare un sentiero di soluzione che io credo oggi abbia portato coloro che sono interessati al problema ad avere le garanzie necessarie che il loro punto di vista potrà essere sostenuto in contraddittorio con l'amministrazione, ripeto, sempre fermo restando che ognuno deve pagare le tasse in relazione alla propria capacità di reddito.

fiscale e psicologico. Da questo punto di vista, quindi, non posso che dichiarare la mia insoddisfazione per la sua risposta alla nostra interpellanza.

ringrazio il senatore Quagliariello che mi offre l'occasione di chiarire in quest'Aula il reale intento del Ministero della solidarietà sociale in merito alla messa in atto di corsi di lingua italiana per gli immigrati. Come sapete, la presenza degli immigrati nel nostro Paese è destinata a crescere e quindi dobbiamo prepararci a confrontarci con la diversità linguistica e culturale tipica delle società multietniche e plurali. Evitare che la convivenza diventi sofferenza, paura e incomprensione è possibile attraverso, anche, l'uso della stessa lingua. Pertanto, riteniamo utile incentivare, dove già esistenti, e creare nuovi corsi di studio della lingua e della cultura italiana su tutto il territorio nazionale, facendo dell'apprendimento della lingua italiana una delle priorità del percorso di integrazione. Infatti, la conoscenza della lingua è il primo strumento di integrazione e di inclusione sociale. Nell'Agenda comune europea per l'integrazione si sottolinea che "la conoscenza di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite sono indispensabili ai fini dell'integrazione e mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione e inclusione sociale". finanziaria di quest'anno ha previsto un fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, al quale è stata assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, sulla cui utilizzazione interverrà il Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità. Allo scopo è in fase di ultimazione una direttiva

misura sul problema dell'immigrazione: il sostegno per l'accesso agli alloggi, l'accoglienza degli alunni stranieri, la tutela dei minori stranieri non accompagnati, la valorizzazione e il supporto alle seconde generazioni, la tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana e dell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto attiene ai corsi di lingua, si è pensato di proporre un progetto di moduli di insegnamento della lingua italiana uguali su tutto il territorio nazionale, in cui l'80 per cento delle ore verrà utilizzato per l'insegnamento vero e proprio della lingua ed il restante 20 per cento di ore per l'insegnamento di elementi di educazione civica di base: la Costituzione italiana, l'ordinamento e le leggi fondamentali dello Stato. Si sta lavorando inoltre con gli enti certificatori riconosciuti - l'Università di Perugia, l'Università Roma Tre, l'Università di Siena e la Società Dante Alighieri di Firenze - perché al termine dei corsi sia possibile ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua raggiunto. La parte del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati destinata ai corsi è di 10 milioni di euro. L'obiettivo è quello di poter attivare corsi per circa 20.000-25.000 studenti. I corsi saranno attuati dalle Regioni attraverso accordi di programma, dagli enti locali e dalle associazioni iscritte nel registro previsto dal Testo unico delle leggi sull'immigrazione, attraverso bandi pubblici. Nella selezione, ovviamente, si privilegeranno quegli enti ed associazioni che hanno una provata esperienza in materia di insegnamento della lingua: si sottolinea che l'iscrizione al registro garantisce la serietà, la qualità e l'affidabilità delle associazioni iscritte. Quindi, da parte nostra, c'è tutta l'intenzione di lavorare in accordo con Regioni, enti locali e associazioni perché questi moduli siano fatti in maniera uguale e con le stesse garanzie dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest. Sono inoltre in via di definizione accordi con la RAI per l'avvio di corsi di italiano che andranno in onda sulla rete pubblica. Infine, si sta lavorando con il Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di programmi di accompagnamento e di insegnamento della lingua italiana rivolti agli alunni stranieri oggi presenti nelle nostre scuole. Tutte queste azioni, dunque, sono progettate con l'obiettivo di dare un grande impulso alla diffusione dell'insegnamento della lingua italiana e di valorizzare quanto si sta facendo in tal senso, attraverso gli accordi di programma con le Regioni e con gli enti locali. Signor Presidente, voglio ringraziare la Sottosegretario per la cortesia della sua risposta.

così come presentato dagli organi di stampa, presentava alcune oscurità e suscitava alcuni dubbi, il primo dei quali si riferiva al fatto che i primi due moduli pilota si sono svolti in due moschee di Roma: la "grande" moschea e quella della Magliana. E poiché in quest'ambito (quello dell'integrazione) anche i luoghi luoghi assumono un valore simbolico e visto che il programma prevede, per l'appunto, non soltanto l'insegnamento della lingua, ma, come è stato correttamente ricordato dalla

noi riteniamo che gli organi dello Stato, i poteri pubblici, debbano compiere un'opera in prima persona se non di iniziativa,

così come scritto in un comunicato del Ministero, vengano favorite associazioni e gruppi di volontariato

l'interrogazione, e che vorremmo assicurare nel prosieguo, è che in questo ambito il controllo sulle

quale motivo, nell'ambito dell'istruzione ordinaria, il maestro della scuola pubblica venga da voi considerato una sorta di sacerdote della cittadinanza, con il compito di trasferire le tavole della legge da generazione a generazione e invece, nel campo dell'immigrazione, che è ancora

associazioni, che molto spesso si ammantano dietro la sigla di associazioni volontarie, si finanziano con denaro pubblico per

in luce un problema importante per il Paese e per il territorio, quello dei Vigili del fuoco di Vicenza. Intanto mi preme sottolineare che la situazione da lui citata non è certo circoscrivibile al solo comando di Vicenza, ma riguarda

Questo è un risultato che si è prodotto anche nel prosieguo del periodo di cui stiamo parlando. La legge finanziaria per il 2007 è servita per pagare una parte di questi debiti.

senatore Zanettin, che riprende le considerazioni del signor Nodari, responsabile della CISL del Veneto, un'attenzione a rilanciare il Corpo e a trovare, insieme, sinergie e soluzioni per lo stesso.

La finanziaria per il 2007 - queste sono risorse che non sono ancora state distribuite ai diversi comandi - ha previsto il finanziamento del settore con un fondo di oltre 60 milioni di euro, derivante dalle entrate straordinarie generate dalle gestioni aeroportuali e dalle addizionali sui biglietti aerei, che servirà per rispondere alle esigenze operative dei comandi italiani. Essendo questo il primo anno, c'è da mettere a regime il finanziamento del fondo,

riflessione con le organizzazioni sindacali per le procedure di stabilizzazione del personale precario. Non mi soffermo su questo punto, ma il senatore Zanettin sa che il Corpo ha al suo interno oltre 10.000 persone che svolgono funzioni

e darà una risposta soprattutto nelle Regioni del Nord, dove più alta è la carenza di organico generata dalla turnazione delle persone che poi, essendo assunte nella pubblica amministrazione, chiedono di tornare a casa. In più, il decreto-legge n.

rispondere alle esigenze di carattere generale. Nello specifico, per quanto riguarda Vicenza, ho già dato indicazione ai nostri uffici di provvedere alle esigenze immediate facendo fronte a bollette i cui debiti non risalgono agli ultimi mesi, ma, ahimè, ad un periodo molto più

persone che entrano in servizio il 19 luglio (quindi, oggi). Inoltre, è in progetto la riqualificazione di tutti i comandi

Regione, ci dovrà essere una corrispondente riqualificazione degli organici e, quindi, una corrispondente risposta organizzativa. In più, colgo l'occasione per dire

stiamo studiando la predisposizione di una bozza di convenzione che mi auguro possa arrivare in tempi rapidi; allo stesso modo, stiamo chiudendo tale intesa con la Regione Lombardia, lo abbiamo già fatto con la Regione Sardegna e la Regione Campania,

compiono nella Provincia di Vicenza circa 6.000 interventi l'anno, mancano infatti - lei l'ha riconosciuto - sia uomini sia mezzi. La nostra Provincia è la terza tra le più industrializzate d'Italia per il numero di addetti, vi sono presenti molte aziende potenzialmente pericolose, in essa insiste un'asse infrastrutturale, tra le più trafficate d'Italia, come l'autostrada A4 Milano-Venezia, interessata molto spesso da gravi incidenti stradali, per questo necessita di un servizio efficiente. Tuttavia, ciò nonostante, il comando dei Vigili del fuoco di Vicenza rischia, come lei ha riconosciuto, signor Sottosegretario, un autentico collasso per carenza di risorse. Nell'anno in corso è stata messa a disposizione per il carburante e la manutenzione degli automezzi la somma di 120.000 euro, del tutto inadeguata, se solo si considera che lo stanziamento per l'anno 2003 era pari a 320.000 euro e all'epoca fu appena sufficiente a far fronte alle necessità. Il Comando ha oggi debiti per bollette Telecom e AIM (acqua, gas e luce) per circa 200.000 euro e, ad oggi, non vi sono risorse per farvi fronte. Anche gli organici sono inadeguati; a fronte di una pianta organica di 272 vigili del fuoco, in realtà gli addetti reali oggi sono soltanto 205 e le squadre di intervento vengono composte anche ricorrendo a due «discontinui», quando la regola ne prevede uno solo. Lo scorso 6 luglio è stata recata a questo prestigioso Corpo la massima umiliazione con l'AIM, società per azioni, ex municipalizzata del Comune di Vicenza, che ha inviato una raccomandata di diffida, con cui ha minacciato il taglio della fornitura del gas metano ove non cessasse immediatamente la morosità. Per fortuna, per intervento del Prefetto, tale eventualità è stata rinviata per qualche settimana, ma il pericolo incombe, anche perché esistono dei tristi precedenti. Abbiamo infatti appreso che nelle scorse settimane il comando dei Vigili del fuoco di Venezia ha subìto proprio l'onta del taglio della fornitura del gas. Nel frattempo, lo stesso ministro Amato, per quanto ci risulta, nel corso di un'audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera, ha candidamente riconosciuto di aver invitato i comandi periferici del Corpo a non pagare le bollette per mancanza di fondi e ad utilizzare quei pochi che ci sono per fare il pieno ai mezzi. Per questo raccolgo con scetticismo le parole che lei, onorevole Sottosegretario, oggi ha pronunciato. I nuovi assunti del Corpo, in realtà, coprono a malapena quelli che nel frattempo si sono trasferiti in altre Regioni. A questo proposito, mi permetterei di invitare il Ministero a considerare il fatto di dare corso a concorsi regionali e non nazionali, in modo da evitare che chi vince magari il concorso, dopo pochi anni, quando maturano i termini di legge, chieda il trasferimento nelle Regioni di origine lasciando scoperte Regioni come il Veneto, nelle quali lei stesso riconosce la sussistenza del fenomeno. La riqualificazione del comando di Vicenza è un progetto del quale si parla da molti anni saremmo molto contenti se ciò avvenisse. Per il momento ci accontentiamo di essere tranquilli che, se le nostre famiglie hanno un problema di sicurezza e chiamano il "115", senza indugio arriva un'autobotte rossa e non ci si sente rispondere che, invece, deve rimanere ferma nell'autorimessa per mancanza di carburante come, ad oggi, stiamo rischiando. Per questo, onorevole Sottosegretario, continueremo ad incalzare il Governo, per mantenere l'attenzione desta sulle problematiche di sicurezza del nostro territorio.

senatori, rispondo all'atto parlamentare in esame, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si precisa che sulla vicenda segnalata nell'atto parlamentare il Ministero della salute ha tempestivamente richiesto notizie in merito all'assessorato alla sanità del Veneto. L'assessorato ha comunicato che da parte dell'azienda ULSS n. 4 «Alto Vicentino» sono state adottate le indicazioni contenute nella «procedura operativa tubercolosi», approvata con delibera regionale n. 866 del 7 dicembre 2005, che comprende anche l'istituzione di un dispensario funzionale per il controllo della malattia tubercolare, in accordo con le linee guida nazionali e regionali. L'intervento si è basato sulla diagnosi tempestiva, sul controllo specialistico di alto livello qualitativo, sull'individuazione e monitoraggio dei contatti, su un trattamento efficace e sul «*follow-up*». Il 29 gennaio 2007 una ragazza di 16 anni, di origine congolese, è stata ricoverata d'urgenza presso l'unità operativa profilassi malattie infettive (UOC) della azienda citata, per sospetta TBC polmonare, a seguito di riscontro anamnestico effettuato su di un fratello convivente ricoverato il giorno precedente presso la stessa unità per TBC bacillifera, in quanto la ragazza presentava sintomatologia analoga a quella del fratello. Dagli esami radiologici, i sanitari rilevavano un'affezione polmonare in atto; pertanto, venivano adottate le precauzioni di isolamento previste per le infezioni a trasmissione aerea, fornendo inoltre alla paziente tutte le informazioni relative alle procedure adottate e ai comportamenti da assumere. Il giorno 30 gennaio 2007, non appena disponibile il referto dell'esame batterioscopico dell'escreato, il direttore dell'unità operativa complessa comunicava telefonicamente l'esito ai medici della sezione malattie infettive del dipartimento di prevenzione, sottolineando anche i dati più rilevanti dal punto di vista epidemiologico, desunti dall'anamnesi della paziente. La TAC, eseguita qualche giorno dopo il ricovero, ha confermato un quadro clinico compatibile con TBC polmonare, come già riscontrato dal laboratorio di microbiologia dell'azienda sanitaria. A seguito del trattamento antibiotico instaurato, c'è stato un graduale e costante miglioramento delle condizioni cliniche della paziente, dimessa il 20 febbraio 2007, dopo 22 giorni di trattamento farmacologico osservato e ben tollerato e dopo un ulteriore esame batterioscopico negativo. In considerazione della buona risposta alla terapia e dell'abbattimento della carica microbica, la paziente è stata affidata alle cure dell'ambulatorio di pneumatologia, presso il quale, fino ad oggi, è sottoposta ai controlli necessari. Il 31 gennaio 2007 anche i familiari dei due giovani hanno effettuato il *test* di *screening*. Per quanto riguarda gli interventi di sanità pubblica effettuati, si precisa che il 30 gennaio 2007, a seguito della segnalazione del direttore della citata unità, il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica (SISP) ha contattato il preside del liceo classico «Giacomo Zanella» di Schio, fornendo le indicazioni previste dalla procedura operativa; è stato concordato, inoltre, che l'informazione agli alunni e ai genitori sarebbe avvenuta con comunicazione scritta consegnata per il tramite della stessa scuola. Inoltre, per escludere eventuali casi secondari, è stato consigliato alle persone rimaste a stretto contatto con la paziente di sottoporsi allo specifico *test*. In caso di esito positivo delle analisi, sarebbe stato necessario effettuare ulteriori accertamenti; in caso contrario, occorreva ripetere il prelievo dopo alcuni mesi per escludere un viraggio del risultato. In particolare, sono state fornite indicazioni sulle modalità di effettuazione del *test* ed è stato richiesto al preside di comunicare i nominativi del personale docente e non docente e degli alunni da sottoporre al prelievo. Le persone coinvolte negli accertamenti sono state invitate a presentarsi presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Schio, dove hanno effettuato il *test*, gratuitamente e senza impegnativa, nei giorni 6 e 7 febbraio 2007; per i minori di 18 anni è stata prevista la presenza di un genitore o l'autorizzazione al prelievo. Stante la temporanea indisponibilità dell'abituale *test* di *screening* denominato «Mantoux», i responsabili dell'unità operativa complessa hanno deciso di utilizzare un altro test *in vitro*, denominato «Quantiferon», risultato più sensibile e specifico di quello abitualmente usato. Pur rispettando le necessarie cautele di riservatezza di fronte a problematiche sanitarie, il personale addetto, nella fattispecie, non ha imposto alcuna regola del silenzio nei confronti delle parti interessate e la disposizione degli studenti rispetto al caso in esame. Dopo il primo *screening*, effettuato su 43 soggetti, i casi positivi sono risultati complessivamente 10. Analoga prassi procedurale ed informativa è stata osservata nei mesi di aprile e maggio 2007, in occasione del secondo controllo. I genitori degli studenti risultati positivi sono stati dapprima contattati telefonicamente, al fine di fornire loro opportune ed utili notizie circa gli esiti degli esami I soggetti riscontrati positivi sono stati invitati ad eseguire l'esame radiografico del torace, una visita specialistica tisiologica, nonché a sottoporsi ad adeguato trattamento chemioprofilattico per un periodo di sei mesi; durante il primo mese gli interessati sono stati monitorati, a distanza di quindici giorni, con esami della funzionalità epatica e sono stati informati singolarmente sul concetto di tubercolosi latente, sulla necessità della profilassi e soprattutto sull'assenza di contagiosità. Le successive visite sono state programmate con cadenza mensile. L'azienda sanitaria, che ha curato anche la pubblicazione di una pagina esplicativa della vicenda su un quotidiano locale, ha sottolineato che nelle varie comunicazioni intercorse con l'istituto scolastico è stato sempre fornito il recapito telefonico dell'unità operativa profilassi malattie infettive e che tale opportunità è stata utilizzata esclusivamente da un solo dipendente della scuola interessata. In data 30 maggio 2007, lo stesso SISP ha inviato una lettera anche ai genitori degli alunni delle classi che avevano utilizzato l'aula della 1a classe del liceo classico, invitandoli a far eseguire ai loro figli il *test* in data 7 giugno 2007; due degli alunni sono risultati positivi. Pertanto, in applicazione del concetto di sorveglianza «a cerchi concentrici», lo *screening* è stato allargato ad ulteriori tre classi e sono stati sottoposti a prelievo altri 66 studenti. Il preside del liceo ha richiesto all'azienda un incontro informativo per illustrare quanto era stato fatto e per tranquillizzare e rassicurare studenti e genitori; infatti nella prima settimana dello scorso mese di giugno sono stati organizzati due incontri pubblici. Deve essere ricordato che il medico specialista di malattie infettive e/o di sanità pubblica riammette i pazienti in comunità solo dopo che è stata accertata, con controlli clinici ripetuti, la mancanza di contagiosità dei soggetti coinvolti, valutando i risultati dei controlli radiologici nel corso del trattamento antitubercolare e la negatività microbiologica dell'esame diretto e della coltura dell'espettorato. L'azienda sanitaria interessata ha confermato che la contagiosità di questa patologia, dopo l'applicazione efficace e tempestiva delle procedure di controllo e dopo una terapia antitubercolare ben monitorata, è negativa, come risulta dal fatto che il micobatterio della tubercolosi non si è diffuso nel liceo di Schio. Per gli aspetti più generali della problematica "tubercolosi", si sottolinea che tale patologia è una malattia infettiva causata da un batterio denominato L'Italia, con meno di 10 casi notificati ogni anno per 100.000 abitanti, fa parte dei Paesi a bassa incidenza. Gli interventi da adottare per la terapia e la gestione dei pazienti affetti da tubercolosi attiva, per l'identificazione, la sorveglianza e il trattamento preventivo dei gruppi a rischio e dei contatti, nonché per la sorveglianza epidemiologica della malattia, sono stati definiti nelle "Linee guida per il controllo della tubercolosi" emanate il dicembre 1998, sulla base di un accordo Stato-Regioni. L'intervento più efficace è rappresentato certamente da una diagnosi tempestiva, da un trattamento terapeutico efficace e dalla ricerca dei contatti avuti dai soggetti colpiti, sia per i cittadini italiani che per gli immigrati. Gli interventi preventivi, svolti in collaborazione con le associazioni di volontariato e con i rappresentanti delle comunità di stranieri presenti nel nostro territorio, devono essere rivolti particolarmente a quei gruppi di immigrati che, a seguito della situazione di disagio sociale di cui, in molti casi, soffrono, sono ad alto rischio per lo sviluppo della malattia. Relativamente agli immigrati, va detto che le misure di *screening* generalizzato della tubercolosi, in assenza di epidemie, non risultano efficaci nel controllo della malattia; lo strumento più efficace, invece, è la disponibilità piena e completa dell'accesso ai servizi sanitari di diagnosi e cura, nonché la continuità nella lunga terapia farmacologica, che può essere facilitata con l'aiuto di mediatori culturali. Tra le azioni prioritarie, individuate dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute, sono previste la promozione di iniziative per supportare l'attenzione al problema tubercolosi nei gruppi a rischio, la prevenzione e il controllo della tubercolosi per le persone immigrate da Paesi ad alta endemia, e per altri gruppi di popolazione ad elevato rischio (ad esempio, persone con infezione HIV). Il Ministero della salute ha elaborato un piano di prevenzione, che è stato sottoposto al parere positivo del coordinamento interregionale per la prevenzione delle malattie infettive; il piano contiene le azioni da intraprendere, in linea con le raccomandazioni internazionali valide per i Paesi a bassa incidenza della malattia tubercolare. Tra queste vanno ricordate la promozione di una maggiore percezione del problema tubercolosi, l'implementazione di programmi efficaci di controllo della tubercolosi, la qualità del sistema di sorveglianza, una migliore assistenza nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con tubercolosi sospetta e accertata, e una maggiore cooperazione internazionale per un controllo globale e capillare della tubercolosi.

che è stata esposta oggi dal Governo, a giudizio dell'interrogante, tende a minimizzare la criticità della situazione sanitaria che si è sviluppata all'interno dell'istituto «Giacomo Zanella» di Schio**,** che invece è stata assai grave ed è anche emblematica della superficialità con cui è stata trattata la questione dall'autorità scolastica. Infatti, alla fine del mese di gennaio scorso sono stati ricoverati per tubercolosi all'ospedale di Schio - lei lo ricordava poc'anzi - due giovani di origine congolese: una ragazza frequentante il liceo classico «Giacomo Zanella» di Schio e suo fratello. Sono stati informati il preside della scuola, nonché solo i genitori degli studenti della classe frequentata dalla ragazza, che sono stati invitati a far eseguire un *test* ai loro figli per diagnosticare un'eventuale tubercolosi latente. A tutti gli interessati è stata prescritta dalle autorità scolastiche e sanitarie la consegna del silenzio e della riservatezza. Al primo controllo sono risultati positivi 9 studenti, che sono stati subito messi in trattamento antibiotico preventivo. Nel mese di maggio sono risultate positive al *test* altre 8 persone, 7 alunni ed un insegnante; a questo punto è scattato l'allarme fra i genitori degli alunni di tutte le altre classi del liceo. Fra i banchi della scuola girava la TBC e nessuno ne parlava, e né l'autorità sanitaria, né l'autorità scolastica si sono premurate di informare adeguatamente alunni ed insegnanti, mentre la notizia serpeggiava fra gli studenti. Un caso, insomma, gestito male: probabilmente prima ha prevalso la psicosi della reticenza, quindi è stata sbagliata completamente la strategia comunicativa, diffondendo la paura. Speriamo che in futuro, nell'approccio a situazioni analoghe, si evitino gli stessi errori. Provo quindi a rivolgere al Governo alcune proposte metodologiche. Punto primo: ormai da tempo viene segnalata la recrudescenza nel nostro Paese di *virus*, che solo pochi anni fa sembravano definitivamente debellati, come la tubercolosi, a causa dell'ingresso nel nostro Paese di cittadini extracomunitari, provenienti da aree geografiche nelle quali le condizioni igieniche sono assai carenti e detti *virus* sono endemici. Ora, a fronte di questo mutato rischio, le autorità sanitarie dovrebbero essere tenute a porre in essere una attenta politica di prevenzione. E questa politica di prevenzione potrà essere attuata soltanto se i soggetti a rischio saranno sottoposti a preventivi accertamenti sanitari, prima dell'ingresso in comunità, come le scuole o i posti di lavoro, o forse sarebbe addirittura opportuno fossero sottoposti ad accertamenti sanitari prima di essere autorizzati a risiedere nel nostro Paese. Lasciamo perdere il buonismo e l'ipocrisia, se in gioco è la salute dei nostri figli e dei nostri concittadini. La salute pubblica è un bene primario che merita la massima tutela. Punto secondo: quando un focolaio di malattie infettivo viene individuato, lasciamo perdere ogni atteggiamento omertoso (che invece è chiaramente emerso nella vicenda di Schio) e teniamo informata senza reticenze l'opinione pubblica, al di là della *privacy* di cui tanto si parla. Ogni padre ed ogni madre hanno diritto di sapere se nella classe o nella scuola frequentata dai propri figli è presente un focolaio di infezione e devono anche essere liberi di adottare ogni conseguente cautela ritenuta opportuna. In particolare, dev'essere autorizzato, se richiesto dai genitori, l'immediato trasferimento del figlio in altro istituto scolastico. Per timore del discredito dell'istituto scolastico e della paralisi delle lezioni, non è accettabile che gli allievi siano esposti, com'è capitato a Schio, anche al minimo rischio sanitario. Punto terzo: i soggetti che sono portatori di *virus* infettivi devono essere isolati con il massimo rigore, soprattutto se possono entrare in contatto con altri ragazzi. Poiché non sono soddisfatto della risposta ricevuta e del giudizio del Governo sulla vicenda, le preannuncio, onorevole Sottosegretario, che intendo ritornare a breve con altri atti di sindacato ispettivo sulla questione della diffusione di malattie infettive nelle scuole e sulle misure adottate dalle autorità sanitarie per prevenire il ripetersi del fenomeno, nella speranza, come ho già detto, che queste mie sollecitazioni evitino il ripetersi di errori analoghi a quelli registrati a Schio.

salute*. Signor Presidente, senatore Domenico Gramazio, in via preliminare si precisa che il Comando dei carabinieri per la tutela della salute (NAS), nell'anno 2006 e nel primo semestre 2007, ha sottoposto a sequestro prodotti della medicina tradizionale cinese, confezionati in varie forme per un totale di 20.567 confezioni. Nell'ambito dell'attività di contrasto posta in essere nello specifico settore segnalato nell'interrogazione parlamentare, si sottolinea che in Italia il controllo della produzione di farmaci è effettuato secondo criteri e metodiche regolari, e ricomprende sia i medicinali «*branded*» che quelli generici.

alle quali sono soggetti i produttori di farmaci e di materie prime farmacologicamente attive. Relativamente ai Paesi terzi, dove possono essere prodotti medicinali e princìpi attivi a rischio, si precisa che il suddetto decreto legislativo ha consentito per questi Paesi la verifica del rispetto delle GMP. Sono state disposte diverse ispezioni, effettuate con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità; va precisato, peraltro, che già antecedentemente alla normativa citata, l'Italia ha partecipato alle ispezioni svolte dalle organizzazioni internazionali. Nella lotta ai farmaci contraffatti, il nostro Paese è certamente all'avanguardia in Europa, poiché ha da tempo avviato una cooperazione ufficiale con l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d'Europa. Desidero, inoltre, sottolineare che dopo l'allarme lanciato dall'OMS, secondo il quale il 10 per cento circa dei farmaci che circolano nel mondo sarebbero contraffatti, nello scorso mese di aprile è stato costituito un tavolo tecnico, che vede la partecipazione dell'AIFA, del Ministero della Salute, dei NAS e dell'Istituto Superiore di Sanità, per 1'adozione delle opportune iniziative di controllo. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati realizzati corsi formativi per gli ispettori che operano sul territorio nazionale e sono state individuate le necessarie procedure. L'AIFA, inoltre, ha designato un coordinatore delle attività anticontraffazione il quale, in collaborazione con i NAS, deve verificare i casi che possono interessare il nostro Paese tramite il collegamento con le organizzazioni internazionali. Tra le attività già in corso coordinate dall'AIFA e relative al territorio nazionale si segnala quella che riguarda il commercio illegale dei medicinali su Internet che costituisce senz'altro una delle principali fonti di diffusione di medicinali di dubbia qualità. A questo riguardo, si comunica che si sta provvedendo ad un campionamento da siti sospetti che fornirà i dati utili per avviare una campagna informativa ai cittadini sui rischi degli acquisti di farmaci da fonti non controllate. Lo scopo della campagna è quello di una corretta ed obiettiva informazione su tali rischi che possono compromettere la salute dei pazienti, senza creare, tuttavia, ingiustificati stati di allarme nella collettività. Ritengo opportuno, inoltre, fornire in questa sede istituzionale ulteriori notizie che testimoniano la costante attenzione e l'impegno concreto da parte del Ministero della salute e dei NAS nell'attività di contrasto contro qualsiasi forma di contraffazione che costituisca pericolo per la salute pubblica; mi riferisco al recente caso dei dentifrici a marchio "Colgate". Il competente Dipartimento del Ministero, facendo seguito alle notizie diffuse nel primo pomeriggio del 6 luglio da un'Agenzia di stampa, relative alla presenza sul mercato spagnolo di dentifrici contraffatti del suddetto marchio risultati tossici per alta concentrazione di dietilenglicole prodotti in Sud-Africa, Camerun e Cina, riferiva al Comando NAS che l'Autorità sanitaria canadese aveva diramato un'allerta concernente il rinvenimento di un ulteriore dentifricio del tipo "Colgate" (presumibilmente contraffatto) risultato contaminato da batteri aerobici altamente patogeni della famiglia *Enterobacteriacee*. Venivano subito attivati i NAS per verificare la presenza in commercio di dentifrici a marchio "Colgate" che, indipendentemente dalle tipologie segnalate, riportassero sulle confezioni indicazioni esclusivamente in lingua straniera e, pertanto, non conformi Il suddetto comando, pertanto, disponeva la ricerca dei dentifrici a marchio "Colgate" privi di indicazioni in lingua italiana e il sequestro del prodotto. In aggiunta alle specifiche tecniche fornite dall'Istituto Superiore nella mattinata del 7 luglio 2007, che prevedevano la composizione del campione in due aliquote da due confezioni ciascuna, i NAS disponevano anche il prelievo di ulteriore aliquota da mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio. Le ricerche dei Reparti dei Carabinieri eseguite nella sola giornata del 7 luglio terminavano con il sequestro amministrativo, nell'ambito di 27 province, di 19.402 dentifrici "Colgate" non conformi. Le verifiche, proseguite nella giornata del 9 luglio e concluse il 12 luglio successivo, consentivano di rinvenire e sequestrare in ambito nazionale presso 121 rivendite un numero complessivo di 623.285 confezioni di dentifricio "Colgate" con etichettatura non conforme. Sulla base del cessato allarme biologico comunicato dal Ministero della Salute nel pomeriggio del 9 luglio 2007 e dei primi responsi analitici ufficializzati il 12 luglio dall'Istituto Superiore di Sanità, che hanno escluso la presenza di dietilenglicole nei prodotti esaminati, si precisa che tra le confezioni di dentifricio poste sotto sequestro amministrativo non figurano le tipologie di prodotto segnalate dalle Autorità spagnole e canadesi. In attesa dei risultati di ulteriori accertamenti mirati a stabilire i canali di commercializzazione impiegati per l'approvvigionamento dei cosmetici sequestrati si può ipotizzare che i dentifrici, ancorché non conformi sul piano amministrativo, siano originali e provenienti da mercato parallelo poiché all'origine destinati ad altre nazioni. Si segnala, inoltre, che gran parte degli importatori e distributori emersi dall'esame della documentazione commerciale hanno sede in Olanda, Irlanda, Sud Africa, Thailandia, Vietnam, Brasile e Repubblica Ceca. Si precisa anche che sono state sequestrate 1.389 confezioni di dentifricio di altri marchi con etichettatura non conforme, presumibilmente di importazione parallela.

il dentifricio contraffatto. Adesso, i Cinesi si sono impratichiti: sanno, quindi, di dover utilizzare marchi e nomi di fama nazionale e internazionale, cioè, non importano in Italia un dentifricio che si chiama «*Cian cion cion*»,

nei riguardi delle forze dell'ordine, ma anche degli ispettori delle ASL, che hanno una competenza specifica per quanto riguarda prodotti che vengono venduti in strutture come i supermercati o,

che si sa che sono possibilmente contraffatti e venduti a prezzi più bassi per far arricchire i ladri che riescono poi a rivenderli a danno della salute dei cittadini che a volte, inconsciamente, cadono nel tranello.

Signor Presidente, senatore Sergio Divina, con riferimento a quanto prospettato dall'atto parlamentare, è necessario fornire alcune precisazioni sulla patologia «tifo». Con il termine «tifo» possono essere indicate diverse forme morbose: il tifo addominale, il tifo esantematico e il tifo epidemico da pulci. Inoltre, esistono i cosiddetti tifi da zecche, ad eziologia generalmente rickettssiale, trasmessi all'uomo attraverso la puntura di zecche infette. Relativamente al tifo addominale, si precisa che la salmonellosi appartiene ad un gruppo di malattie che vengono trasmesse per via fecale-orale, tramite l'ingestione di alimenti o di acque contaminate da feci di soggetti che hanno contratto la malattia o attraverso animali infetti. può essere compresa nel novero delle «zoonosi», ossia di quelle malattie che possono essere trasmesse naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo. I casi di salmonellosi, che come tutte le zoonosi sono sottoposti a notifica obbligatoria, sono soggetti a sorveglianza tramite Le misure di sorveglianza, prevenzione e controllo delle zoonosi sono state definite nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, secondo il quale le Regioni e le Province autonome provvedono alla sorveglianza dei casi di zoonosi tramite la raccolta e l'analisi dei dati. Tali dati devono essere inviati al Ministero della salute che opera in stretta collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali e con la Commissione europea. L'Organizzazione mondiale della sanità, sul proprio sito Internet dedicato alle informazioni sui focolai epidemici ha riportato frequenti aggiornamenti su casi sporadici di infezione umana da *virus* dell'influenza aviaria verificatisi in Cina; non ha, invece, dato alcuna notizia su presunte epidemie di tifo, di qualunque eziologia, a Shanghai o in altre città della Cina. Anche nell'Outbreak Verification List, attraverso il quale l'OMS invia ad un limitato numero di professionisti della sanità pubblica specifiche informazioni su epidemie di malattie infettive o su altri eventi degni di nota sotto il profilo della profilassi internazionale, non viene mai fatta menzione di focolai di febbre tifoide in Cina. Il sito Internet Promed, che è un sito gestito dalla Società internazionale per le malattie infettive, recentemente fa menzione di una «malattia non diagnosticata dei suini», con molti casi tra i suini domestici e di allevamento, senza, peraltro, riportare casi diagnosticati nell'uomo; negli anni passati, sempre tra i suini, si erano verificate epidemie dovute a *Streptococcus suis*, che occasionalmente avevano provocato anche alcuni casi tra persone che vi erano esposte per motivi di lavoro. Il tifo addominale è, peraltro, una malattia prevenibile con vaccini efficaci, la cui disponibilità è ampia in tutti i Paesi sviluppati. Non appaiono giustificati quindi i motivi di apprensione sul possibile verificarsi in altri Paesi di una malattia che, sotto forma di casi sporadici, continua a manifestarsi anche in Italia e sulla quale l'OMS non ha ritenuto di dover fare alcuna segnalazione ai sensi del Regolamento sanitario internazionale. Si sottolinea, inoltre, che quei viaggiatori italiani, che si recano all'estero in zone endemo/epidemiche per tifo addominale (praticamente gran parte dell'Africa, dell'Asia e dell'America centro-meridionale) che si rivolgono agli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della salute o ai centri autorizzati per le vaccinazioni internazionali, ricevono le necessarie informazioni, e, ove necessario, la vaccinazione antitifica. Sul sito del Ministero, nella sezione dedicata alle informazioni per i viaggiatori internazionali è disponibile una scheda informativa sul tifo addominale, che indica le modalità di diffusione dell'infezione e le misure preventive, concentrate, oltre che sulla vaccinazione, sull'osservanza di semplicissime regole di igiene personale e degli alimenti. Nel caso, meno probabile, che il «tifo» segnalato nell'interrogazione parlamentare, possa essere una delle forme di tifo esantematico, o tifo murino o da zecche, i motivi di preoccupazione dovrebbero essere ancora minori, in quanto si tratta di malattie che si presentano in forma endemica soltanto in particolari condizioni di degrado sanitario; non è un caso che gli ultimi focolai di queste malattie, segnalati in Europa, risalgano al periodo della Seconda guerra mondiale, e che quelli più recenti hanno colpito i campi dei rifugiati in Africa. Per ciò che concerne i vari tipi di "tifo da zecche", questi si presentano solo sotto forma di episodi sporadici, legati alla frequentazione di particolari ambiti (ad esempio, boscaglie), nei quali le zecche trovano il proprio *habitat* ideale. Anche per le malattie trasmesse da zecche, per le quali generalmente non esistono vaccini efficaci, sul sito del Ministero della salute è riportata la circolare n. 10, del 13 luglio 2000, con indicazioni sulle misure di profilassi comportamentale, utili ad evitare la puntura di zecche. Pertanto, sulla base delle misure di sorveglianza attuate e dell'assenza di segnalazioni di allerta epidemica da parte dell'OMS, e a fronte dello *standard* igienico-sanitario raggiunto dal nostro Paese, si può confermare che il rischio di contagio di massa a seguito di scambi commerciali e di movimenti turistici tra l'Italia e la Cina è estremamente basso. Desidero segnalare, infine, che questa Amministrazione ha finanziato un progetto di ricerca a favore del citato istituto e di alcuni istituti zooprofilattici dal titolo «Sorveglianza delle zoonosi in ambito veterinario e integrazione con le attività esistenti in ambito medico ZOONOSI MED-VET»

chi ha presentato questa interrogazione. Al di là del fatto che lei ci ha fatto un'elencazione dei tipi di tifo (rispetto ai quali oggettivamente non possiamo entrare nel merito),

strano che un Governo al quale partecipa tutta la sinistra dell'arco costituzionale (dai pacifisti ai *no global* in poi) possa permettersi di contravvenire proprio su un fronte di grande sforzo

Un'industria multinazionale americana, ma che ha distretti industriali in Europa e anche in Italia, ha richiamato tutta la parte dirigenziale, il *management*,

Non è che questo tranquillizzi proprio tanto. Non vorremmo lanciare allarmismi ingiustificati, ma avremmo voluto avere almeno rassicurazioni forti che purtroppo non abbiamo avuto,

Mi è capitato recentemente di aver visto un volantino che viene distribuito nell'Ospedale di Civitavecchia con cui si invita la popolazione a non bere l'acqua potabile per l'alta presenza di arsenico.

per l'inserimento del genere *Corallium* in Appendice II della Convenzione di Washington (CITES), menzionato nell'interrogazione di cui trattasi, si desidera precisare che il processo di inserimento nelle Appendici CITES non prevede la stipula di ulteriori accordi internazionali e che il suddetto processo di appoggio per l'inserimento di specie nelle Appendici della Convenzione non può essere stabilito dai singoli Stati membri, ma deve essere concordato in ambito comunitario. La proposta per l'inserimento del corallo in Appendice II, avanzata dagli Stati Uniti sulla base di una serie di considerazioni scientifiche, è stata preliminarmente discussa ed approvata in sede di Comitato I della Conferenza delle Parti CITES CITES il 13 giugno. La problematica in questione, in considerazione della rilevanza che essa riveste per le aziende e sulla base di un documento elaborato dalla FAO, che muove da analisi scientifiche diverse da quelle rappresentate dagli USA, è stata oggetto di esame da parte dei Dicasteri interessati interessati (affari esteri, ambiente e tutela del territorio e del mare, politiche agricole, alimentari e forestali, commercio internazionale) con l'obiettivo di approfondire tutti gli aspetti, comprese le ricadute economiche per il settore, dell'eventuale inclusione nella CITES del corallo mediterraneo e di orientare la posizione comunitaria in senso favorevole alla richiesta italiana. In vista della 14a Conferenza delle Parti, la questione è stata dibattuta successivamente anche in seno al Gruppo ambientale internazionale CITES che ha concordato di assumere una posizione ufficiale UE negoziale, basata sulla necessità di approfondimenti ulteriori, e specifici per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, della proposta statunitense e, quindi, sulla concreta applicabilità ed efficacia delle misure di tutela previste. In conclusione, il gruppo ambientale internazionale CITES ha concordato circa l'opportunità di avviare contatti bilaterali sia con gli Stati Uniti, che con altri Stati membri della Conferenza delle parti, al fine di trovare una condivisa soluzione negoziale. Successivamente, in sede di riunione plenaria, il 15 giugno, la Conferenza delle parti CITES ha deliberato di non procedere all'inclusione di tutto il genere *Corallium* in Appendice II, approvando solamente la decisione che prevede l'organizzazione di due *workshop* tecnico-scientifici per un ulteriore approfondimento dello *status* di conservazione del genere da tenersi nel Mediterraneo e nel Pacifico entro la fine del 2008.

credo che il problema sia stato soltanto spostato al 2008, dopo che le Commissioni avranno proceduto a rilevare scientificamente quale sia la situazione del *corallium rubrum* nel Mediterraneo.

quale chiede di sapere quali siano i motivi della ritardata erogazione dello stanziamento previsto in favore del Comune di Rose (CS) nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 maggio 2006, che ha approvato il 13° Programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico e quali siano i tempi previsti per corrispondere la somma stanziata destinata ad opere di messa in sicurezza del territorio, si rappresenta, innanzitutto, che il decreto predetto, per trovare il proprio perfezionamento, doveva essere registrato alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio. Proprio tale Ufficio ha restituito il provvedimento in questione, rilevando la mancata copertura finanziaria del programma nel suo complesso e l'assenza di qualsiasi elemento istruttorio di analisi e valutazione riferito ai progetti ammessi a finanziamento. Inoltre, la lista allegata al decreto si era limitata ad un mero elenco di Comuni con relativo importo finanziato, mancando ogni riferimento all'oggetto dell'intervento. Per i motivi sopra esposti, lo stesso Ufficio centrale del bilancio non ha ritenuto di inviare il decreto alla Corte dei conti per la registrazione. Dal momento, quindi, che la predetta registrazione alla Corte dei conti non è mai avvenuta, il provvedimento in questione non ha mai esplicato la sua efficacia. In ogni caso, le risorse per le politiche di difesa del suolo per l'anno 2006 sono state rese disponibili, a seguito della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia del 3 maggio 2006, notificato alla Direzione generale per la difesa del suolo con nota dell'8 maggio 2006. La Direzione generale per la difesa del suolo, a seguito della citata comunicazione delle risorse disponibili per gli interventi di difesa del suolo per l'annualità 2006, ha provveduto ad attivare la procedura prevista dal comma 432 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che prevede che il Ministro, d'intesa con le Regioni o gli enti locali, individui il programma di interventi urgenti per la rimozione del rischio idrogeologico. Si segnala che il Ministro ha richiesto esplicitamente, attraverso il proprio Ufficio di gabinetto, alla Direzione generale per la difesa del suolo che tale programma fosse predisposto d'intesa con le Regioni. Ciò anche per garantire l'individuazione di interventi di reale priorità e urgenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sul rischio idrogeologico approvati su tutto il territorio nazionale e predisposti dalle Regioni e dalle Autorità di bacino. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2006 (registro n. 6, foglio n. 325), è stato così approvato, con l'intesa formale delle Regioni su tutti gli interventi individuati, il piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, costituito da n. 311 interventi per un importo di circa 220 milioni di euro, tra i quali non rientra il finanziamento oggetto della presente interrogazione. Tali risorse messe in campo, per quanto esigue rispetto agli oltre 1.600 interventi proposti

e ancora più esigue rispetto alla cifra necessaria per la sistemazione dei bacini su tutto il territorio nazionale, stimata in circa 40 miliardi di euro, consentono comunque di attivare 311 cantieri sul territorio nazionale. La Direzione generale per la difesa del suolo ha inoltre già provveduto a impegnare l'intera somma e contemporaneamente a erogare agli enti attuatori risorse pari a oltre il 90 per cento del totale impegnato.

Tuttavia, la richiesta di fondi per il riassetto territoriale di questo nostro Paese è stata avanzata e abbiamo risorse, anche quest'anno, da mettere in

giunge a proposito e consente di dare una risposta a tutti i Comuni che hanno queste necessità, perché si adoperino a presentare istanze documentate in maniera adeguata per poter consentire al Ministero una lettura ed un

gettando migliaia di famiglie in mezzo alla strada, distruggendo l'intera economia locale, provocando morti e feriti. Un anno fa,

seria battaglia all'interno della mia coalizione per ottenere qualcosa per i tre paesi distrutti, cioè lo

ma ai circa 70 e più paesi calabresi che erano evidenziati già nel decreto Matteoli e che sono ancora